Onorevoli colleghi, lo scorso 19 giugno - stroncato da un malore al termine di un intervento a un convegno giuridico è improvvisamente scomparso Pietro Milio, nostro collega senatore della XIII legislatura. Penalista tra i più illustri del foro di Palermo, era nato a Capo d'Orlando 66 anni fa: la sua cultura profondamente liberale ne informava l'impegno pubblico e la riflessione giuridica, donando alla sua attività professionale il profilo di un garantismo autentico, ben al di là di quanto imposto ad un avvocato dai doveri d'ufficio. La sua attività processuale era caratterizzata da un rigoroso rispetto delle regole e delle procedure, pervicacemente perseguito in tutti gli atti da lui compiuti e, di conseguenza, preteso con forza e determinazione da tutte le controparti, nella ferma convinzione che, in un contesto di tale rilevanza per la sua capacità di incidere sulle libertà individuali, quale quello della procedura penale, il rispetto delle forme non fosse mai del tutto scindibile dalla difesa nel merito. Protagonista, nel suo ruolo di difensore, di alcuni tra i più importanti processi celebrati a Palermo negli ultimi anni, fu strenuo sostenitore della lotta alla mafia. Era sua convinzione, però, che la lotta alla criminalità organizzata andasse condotta, in primo luogo, attraverso un sapiente e tenace utilizzo dei metodi investigativi tradizionali, piuttosto che attraverso il ricorso - da lui ritenuto spesso eccessivo e privo di adeguate garanzie - alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A sostegno delle sue tesi Pietro Milio era solito richiamare il metodo istruttorio di Giovanni Falcone, che non rifiutava affatto il ricorso allo strumento dei collaboratori di giustizia, ma sottoponeva le loro dichiarazioni ad uno stringente riscontro investigativo non soltanto prima di qualsiasi utilizzo processuale, ma anche prima di qualsiasi divulgazione pubblica delle informazioni ricevute. Eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nelle liste del Patto Segni, nella XII legislatura, passò in seguito con la Lista Pannella, ritenendo quella collocazione più compatibile con la sua cultura laica e liberale, ed in occasione delle elezioni del 1996 entrò a far parte di questa Assemblea, unico eletto nelle file radicali. Membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione giustizia, fu relatore di importanti disegni di legge in materia giudiziaria e penale, tra cui, in particolare, quelli che condussero all'approvazione della legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, e della legge 8 marzo 2001, n. 40, in materia di tutela del rapporto tra le detenuti madri ed i loro figli minori. Anche al termine dell'esperienza parlamentare, Pietro Milio aveva continuato a svolgere un'intensa attività politica all'interno dell'area culturale laica e liberale, nel generoso tentativo di giungere al coordinamento ed all'unificazione delle diverse realtà politiche che fanno riferimento a questa identità. Con la sua improvvisa scomparsa perdiamo tutti un raffinato giurista, un grande avvocato, un sincero garantista e - mi si consenta - un caro amico personale: ciò rende la nostra riflessione pubblica sui diritti e sulle garanzie, sulla laicità e sulla giustizia inevitabilmente più povera. Nella certezza dell'insopprimibile forza della testimonianza di chi, come Pietro Milio, non ha mai rinunciato a manifestare con coraggio, anche contro l'opinione dominante, la forza delle proprie idee sulla libertà e sulla giustizia, invito tutti i colleghi ad osservare, in sua memoria, un minuto di silenzio e di raccoglimento.

attento e combattivo, in Aula come nella Commissione giustizia del Senato, Pietro Milio ha sempre mostrato particolare garbo nei confronti di tutti, con i quali amava chiacchierare con le sue buone maniere di gentiluomo siciliano. Eletto alla Camera nel 1994 tra le file del Patto per l'Italia, prima di quella elezione aveva militato nel Partito Liberale Italiano e, dopo l'esperienza con Segni, nel Partito Radicale: un'attività, quella all'interno del partito di Marco Pannella, che l'ha visto accedere a Palazzo Madama due anni più tardi. Coloro che l'hanno conosciuto ricordano inoltre, accanto alla sua opera come brillante avvocato e giurista, un merito particolare: l'aver presentato, il 25 giugno 1997, l'unica interrogazione sull'affare Telekom Serbia, a ridosso della conclusione di quel discutibile accordo che comportò, in cambio dell'acquisto da parte di Telecom Italia (allora controllata dal Ministero del tesoro) del 29 per cento di Telekom Serbia, il versamento di oltre 450 milioni di euro dei cittadini italiani direttamente sui conti correnti di Slobodan Milosevic, soggetto contro cui, solamente 22 mesi più tardi, l'Italia sarebbe intervenuta militarmente. L'interrogazione all'epoca era diretta al presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, e al ministro delle poste e telecomunicazioni, Antonio Maccanico. Inutile dire che la risposta non è mai arrivata. Nella sua vita professionale, come in quella politica, ha avuto sempre a cuore la verità ed ha rifuggito sempre dalle voci di palazzo non suffragate da prove certe, come quelle sulle vicende giudiziarie del generale Mori e del colonnello Di Caprio. Una vita controcorrente, la sua, che lo ha portato a difendere le proprie idee e i propri assistiti con impegno, passione e fervore. Un uomo, un politico, un professionista, la cui voce arguta ed appassionata mancherà al dibattito politico del nostro Paese.

innanzitutto la voglio ringraziare per le parole che ha voluto usare nel ricordo del nostro collega Piero Milio.

anche delle sintonie di approccio alla politica, che temo si stiano perdendo: sarebbe

che ha connotato la vita politica di Piero Milio. Lei ha ricordato che Piero arriva a una militanza politica attraverso il Partito Liberale.

Palermo, anticipatori - mi consentano i colleghi - di tante vicende drammaticamente attuali - temo - del nostro Paese, indicatori di quel tanto che si agita nel sottobosco della politica e dell'amministrazione anche oggi, facendo strame di ogni norma costituzionale e di legge. Era un liberale d'altri tempi, si dirà: c'è da augurarsi che siano i tempi futuri, perché davvero ne avremmo, noi e le istituzioni, un grande bisogno.

ma che è molto importante. Piero Milio si appassionò alla situazione drammatica e illegale dei manicomi criminali.

Scrisse un buon disegno di legge, una proposta praticabile che poneva l'accento sull'aspetto sanitario di quelle strutture. In Parlamento ne sono stati depositati solo due (forse dovremmo andare a riprenderli) il suo e quello scritto dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Questo volevo aggiungere brevemente agli

però, questa sua capacità di credere nella giustizia, di credere alle procedure, non a quelle spettacolari ma a quelle sostanziali,

se è vero, come diceva Manzoni, che talvolta il buon senso si nasconde per paura del senso comune, bisogna dire che il buon senso che ispirava la vita e l'attività, prima civile e poi politica, di Piero Milio non si nascose mai e mai fu travolto dal fu travolto dal conformismo dei tempi, né dall'ipocrisia del politicamente corretto. La sua esperienza umana e professionale, i suoi modi da signore d'altri tempi, come altri colleghi hanno detto, la sua passione lasciano, in chi, come il sottoscritto, ha avuto il privilegio di conoscerlo e di essergli amico, una traccia indelebile e più di un insegnamento, soprattutto in materia di reale di reale esercizio e godimento dei diritti umani. Piero Milio era un uomo libero, leale, onesto, impegnato, convinto e consapevole del fatto che il suo compito di uomo non potesse essere legato soltanto agli aspetti privati, familiari e personali, ma dovesse essere rivolto anche alla società nella quale egli viveva, al nostro Paese, alla Sicilia, al mondo della giustizia, ai più deboli. Piero Milio è stato senatore della Repubblica nella legislatura 1996 2001, unico rappresentante della Lista Pannella, anche grazie alla mancata presentazione, nel suo collegio, di una candidatura del centrodestra. Egli non aveva una storia di militanza radicale, ma esercitò il suo mandato con impegno e lealtà nei confronti dei radicali, condividendone le scelte civili. Era - come dicevo - un convinto liberale, e in tal senso si battè per la difesa dei diritti umani, dei più deboli, della giustizia giusta, non mettendo mai davanti a sé né pregiudizi né preconcetti, anche quando questo poteva sembrare fuori moda. Anzi, soprattutto, quando questo sembrava fuori moda. Da professionista, fu tra i primi a rompere il silenzio dell'avvocatura contro la mafia e ad assumere le parti civili dei familiari, spesso isolati da azzeccagarbugli in cerca di parcelle e non di verità e di legalità. Ma Piero Milio fu precursore anche di associazioni come «Addio Pizzo» ed altre che si battevano per liberare la Sicilia dall'oppressione mafiosa. Piero Milio, però, non fu mai vicino a certa antimafia conformista che vedeva la repressione quale unico strumento di lotta a Cosa nostra. Ricordo con lui innumerevoli incontri che riguardavano la struttura delle carceri, persino la struttura della pena;

non esitò a criticare il regime del 41-*bis* per i suoi aspetti particolarmente duri. In conformità con le sue idee, nel 1997, fu l'unico parlamentare ad interrogare senza esito il Governo Prodi sull'*affaire* Telecom Serbia e sui contributi italiani a Slobodan Milošević, nonostante l'embargo internazionale che in quel momento era in vigore contro Belgrado. Nel corso della sua attività parlamentare fu relatore alla Commissione giustizia del Senato del disegno di legge sulla modifica al codice di procedura civile, in tema di competenza territoriale, per le cause promosse da o contro magistrati e del disegno di legge riguardante misure alternative alla detenzione, a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Prima di sedere in quest'Aula, Piero Milio era stato deputato nazionale, eletto nelle liste del Patto Segni, distinguendosi sempre per la sua attività in difesa dei diritti umani e civili. questo ricordo di Piero Milio ribadendo il suo impegno per una giustizia giusta, per pene e carceri non afflittive, bensì in grado di recuperare alla legalità quanti hanno violato la legge, e per una società più libera, liberale e tollerante, nel pieno rispetto dei contenuti dell'articolo 27 della Costituzione. Come dimenticare, a tal proposito, le sue battaglie in favore di processi trasparenti e di giudizi fondati su fatti e prove e non su teoremi o soltanto su pentiti rivelatisi per per nulla tali? Egli credeva nel suo impegno, con il quale sfidava, ogni giorno, la sua fragile salute che, all'età di 66 anni, lo ha prematuramente tradito nel pieno della sua attività, alla fine di un convegno, privando il nostro Paese di un uomo che, pur non essendo per nulla incline a qualsiasi protagonismo, è stato un grande protagonista della storia di questo Paese. Alla famiglia di Piero Milio giungano le espressioni di cordoglio di tutto il Gruppo del Popolo della Libertà e mie personali.

bisogna subito ricordare che il provvedimento che ci accingiamo ad affrontare nell'Assemblea del Senato nasce da un'esigenza specifica, quella di rispondere in maniera efficace alle pressioni crescenti dei mercati, generate dall'emergere di un significativo *deficit* *deficit* dei conti pubblici della Grecia. Si è data così una sorta di attuazione anticipata all'intento comune, espresso in sede europea dalla Commissione, finalizzato a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, preso il 12 maggio scorso, e contestuale alla creazione di un meccanismo di stabilizzazione deciso e attuato in sede europea. È evidente che la situazione dei conti pubblici in Europa sta determinando un processo di concentrazione delle politiche finanziarie a livello sovranazionale. Seppure comprensibile, dati gli elevati livelli di debito di alcuni Paesi membri, tuttavia questo processo, ad oggi, non è privo di criticità e rischia di creare alcune contraddizioni, se insieme ad esso, in particolare, non vengono rafforzate la sovranità e la rappresentatività democratica delle istituzioni europee. Su questi aspetti, occorre svolgere un'attenta riflessione. Il coordinamento degli interventi di politica economica e finanziaria potrebbe portare, molto probabilmente già dal prossimo anno, alla fissazione dei principali aggregati dei bilanci nazionali da parte delle istituzioni europee. È evidente che si tratterà di una ulteriore cessione di quote di sovranità nazionale alle istituzioni europee ovviamente, al fine di rendere più cogenti questi strumenti di controllo della spesa, sarà necessario - lo ribadisco un contestuale processo di miglioramento della *governance* politica europea, in particolare della sua democraticità. Anche in questa chiave la manovra di bilancio in esame, pur anticipata rispetto alle scadenze usuali, è intesa a ridurre l'incertezza per gli operatori economici e rende evidente che la politica di bilancio è al momento fermamente orientata a raggiungere gli obiettivi indicati. La manovra, che ha un impatto a regime quantificato circa l'1,5 per cento del prodotto interno lordo, è destinata pertanto prevalentemente a correggere l'andamento dei saldi riportandoli in linea con il percorso di riduzione del*deficit* tracciato nei documenti di bilancio in sede pluriennale. Rispetto all'andamento del ciclo economico, la manovra si colloca nella fase di consolidamento della ripresa ma bisogna tener presente che la crisi del biennio 2008‑2009 non ha ancora esaurito i suoi effetti sia sull'economia reale sia sulla finanza pubblica. Nel complesso, l'entità della correzione - che, voglio ricordare, è rimasta intatta nel corso dell'esame in Commissione bilancio è da ritenersi adeguata a raggiungere gli obiettivi di indebitamento netto nel quadro macroeconomico. Il Governo, nel corso dell'esame in Commissione, ha evidenziato l'impatto sulle variabili macroeconomiche, La grande questione che si è posta nella discussione in Commissione è cioè l'effetto della manovra sia recessivo, e quindi contrastante con la necessità di aiutare la ripresa in corso. In realtà, i documenti hanno mostrato che non vi è dubbio che una manovra da 25 miliardi ha un limitatissimo effetto, effetto, non recessivo ma di minor crescita, quantificata in frazioni, in decimali di punto, ma è evidente che ad essa è anche associato un effetto di contenimento dei costi pubblici che, senza dubbio, un effetto di sviluppo non quantificabile al momento ma che, ad avviso del Governo, sarà apprezzabile e probabilmente superiore agli effetti recessivi in senso stretto del contenimento dei conti pubblici. A tale proposito, va ricordato che la manovra è basata in larga misura su riduzioni della spesa corrente oltre che su misure di contrasto all'evasione. Tale composizione degli interventi appare complessivamente appropriata, considerata in particolare la dinamica divergente che hanno registrato rispettivamente la crescita economica e la spesa corrente nell'ultimo decennio a motivo dei diversi determinanti dei due aggregati: si è cioè visto che nel corso del decennio all'aumento del *deficit* e del debito è corrisposta una diminuzione della crescita economica. Dunque, vale ciò che ho detto prima: certamente, ad una riduzione del debito e del *deficit* corrisponde un significativo contributo alla crescita, al di là degli effetti immediati che una manovra può avere. Sul versante della spesa le scelte fatte, in massima parte obbligate, corrispondono pertanto alle numerose evidenze teoriche e empiriche, che suggeriscono come la riduzione della spesa pubblica, in particolare nei Paesi con condizioni di finanza pubblica particolarmente difficili, precostituisca le condizioni della crescita economica. Voglio dire a tutti che è vero che talvolta si portano ad esempio le esperienze di altri Paesi, che certamente bisogna far tesoro delle esperienze di altri Paesi, ma non v'è dubbio che le le manovre economiche e finanziarie di ciascun Paese devono poi tener conto delle condizioni specifiche di quel Paese, e noi sappiamo che il nostro è un debito pubblico assolutamente rilevante nel contesto dei Paesi occidentali. Il peso del debito pubblico - dicevo - impone infatti una riduzione dello stesso. Per quanto riguarda la manovra, nel dettaglio, gli interventi per più del 70 per cento sono rappresentati da riduzioni lineari nelle spese dei Ministeri e da riduzioni dei trasferimenti a Regioni ed enti locali. Per comprendere meglio le decisioni, per quanto concerne il comparto del pubblico impiego va segnalato che in quest'ultimo decennio la dinamica delle retribuzioni in questo comparto ha visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello di altri comparti. In tale direzione, una parte significativa delle misure riguarda anche la finanza decentrata. Anche in questo caso si interviene su un settore che, nel suo complesso, ha evidenziato negli anni un andamento della spesa divergente rispetto al PIL. L'esame in Commissione del provvedimento è stato intenso ed impegnativo. Come è noto, si è reso necessario chiedere più proroghe del termine inizialmente fissato. Ciò è stato necessario, in particolare, per tener fede all'impegno preso con tutte le parti politiche di esaminare tutti gli argomenti nella sede più propria della Commissione. E così è stato. Ho inteso rispettare questo impegno, naturalmente in accordo con la Presidenza del Senato, per evitare il rischio di uno svuotamento sostanziale dell'esame del provvedimento nel Senato della Repubblica, soprattutto nell'ipotesi in cui il Governo dovesse ritenere necessario ricorrere al voto di fiducia in relazione ai tempi stringenti per la conversione del provvedimento. Si può cioè dire che la manovra di bilancio è stata attentamente discussa, esaminata ed approvata nelle Aule parlamentari, nella fattispecie, nell'Aula della Commissione bilancio. Nel corso dell'esame in Commissione, infatti, sono state approvate numerose modifiche. Mi limiterò, naturalmente, alle più importanti, si possono suddividere sostanzialmente in quattro principali capitoli: previdenza, enti locali, pubblica amministrazione ed entrate. In materia previdenziale, purtroppo - mi si consenta una riflessione - l'emendamento presentato, che costituisce una stabilizzazione di lungo periodo dei conti pubblici, è stato evidenziato sulla stampa per una piccola questione, peraltro immediatamente espunta in Commissione. Non si è ragionato - ed è invece utile farlo - sulla portata strutturale di questo emendamento. In materia previdenziale, infatti, è stato previsto l'innalzamento dei requisiti anagrafici in rapporto all'allungamento della speranza di vita accertato dall'ISTAT, in modo da incrementare i predetti requisiti in misura pari a tale aumento. Viene data attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea elevando a 65 anni, a decorrere dal 2012, l'età per il pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti della pubblica amministrazione. Vengono poi apportate modifiche alla norma sulla ricongiunzione pensionistica con finalità di armonizzazione e razionalizzazione; viene previsto anche per il 2010 l'utilizzo delle somme rivenienti dai contributi dei datori di lavoro pubblici alle forme pensionistiche complementari al fine di avviare i fondi pensione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Insomma, una riforma strutturale che certamente è un punto fermo nella stabilizzazione di medio-lungo periodo dei conti pubblici. In materia di invalidità civile, la Commissione ha approvato una correzione assai significativa del testo del provvedimento. mantenuta la percentuale di invalidità al 74 per cento oltre la quale scattano una serie di benefici per gli invalidi.

un notevole miglioramento delle norme per il contrasto alle false invalidità e per il controllo delle invalidità al fine di evitare il ricorso

In questa chiave si propone un più ampio coinvolgimento, anche in sostituzione, dell'INPS nell'ambito del processo di accertamento delle condizioni Con riferimento al comparto Regioni-enti locali, oggetto di un'importante discussione a livello nazionale, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella determinazione delle riduzioni dei trasferimenti da praticare nei confronti dei predetti enti territoriali. In sostanza, la modifica centrale apportata è stata nel senso di dare alle Regioni e agli enti flessibilità e autonomia nel fissare i comparti e le modalità per rispettare la fissazione dei saldi, che invece è rimasta invariata. Importanti agevolazioni ai fini del patto di stabilità sono state concesse ai Comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto e per gli enti per i quali, negli anni 2007-2009, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali. Sempre con riferimento al comparto enti locali viene istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, finalizzato ad agevolare i termini di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Viene soppressa l'agenzia autonoma per l'adesione all'albo dei segretari comunali e provinciali e vengono trasferite le relative risorse e funzioni al Ministero dell'interno. Di conseguenza, viene soppresso il contributo a carico delle amministrazioni comunali e provinciali, compensato con una riduzione del contributo ordinario

Ulteriori novità riguardano i crediti maturati nei confronti degli enti territoriali dal Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti. A partire dal 1° gennaio 2011, tali crediti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo. Se gli enti citati non dovessero versare l'importo del credito certificato entro i termini stabiliti all'agente della riscossione, si procederà alla riscossione coattiva nei confronti degli enti stessi. Non è ciò che

Ci auguriamo che, compatibilmente con il contenimento a regime dei conti pubblici, si possa di nuovo mettere mano ad un problema vero,

Sono state chiarite alcune questioni ed alcuni aspetti procedurali relativi al Comune di Roma. della pubblica amministrazione e in particolare della riduzione dei costi degli apparati amministrativi, sono state apportate alcune correzioni per tenere conto in particolare delle peculiarità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È previsto, inoltre, che le economie derivanti dal piano di consegna dei mezzi e sistemi d'arma, nonché derivanti dal canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa siano finalizzate alle esigenze del Ministero della difesa.

delle procedure di bilancio relative alla consegna dei sistemi d'arma, mettendo al riparo il bilancio dello Stato da ogni possibile problema. Siamo sempre disponibili a fare ancora meglio, ma la discussione su questo punto è stata di particolare rilievo e mi pare giusto sottolinearlo. Si è proceduto anche alla sistemazione delle norme afferenti alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, rendendo le disposizioni meno stringenti nei confronti di determinate istituzioni e, in particolare, delle agenzie fiscali. Si segnala ancora, nell'ambito del comparto sicurezza-difesa, l'istituzione di un fondo di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011-2012 destinato alle esigenze del personale adibito alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al soccorso pubblico. Per il personale della magistratura, a fronte del venir meno di una serie di misure volte a contenere il trattamento economico, si procede nel periodo 2011-2013 alla riduzione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 3 della legge 19 27, percepita dal medesimo personale. Forse una più attenta lettura degli emendamenti nel corso dei fine settimana avrebbe portato ad una migliore conoscenza di quanto è stato fatto nei confronti di questi comparti.

Un'altra rilevante modifica apportata in Commissione riguarda la disposizione volta ad utilizzare le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP 6 del 1992 relative alle fonti rinnovabili, inclusi i certificati verdi, in favore di interventi nel settore della ricerca e dell'università. Sempre in tema di certificati verdi, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del Gestore servizi energetici (GSE), dei certificati verdi, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso. In materia fiscale sono state introdotte modifiche in tema di fondi immobiliari. È prevista, inoltre, una stretta sui fondi immobiliari "veicolo", circoscrivendo la vigilanza della Banca d'Italia e il regime fiscale solo ai fondi che gestiscono risparmio diffuso. Sono stati amplificati gli scopi e gli obiettivi connessi alle cosiddette reti di impresa, prevedendo altresì la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune con una particolare disciplina fiscale.

complessa, anche sotto profili di rilevanza costituzionale: quella relativa all'immediata esecutività dell'accertamento, che ora non c'è più. Il termine è stato spostato a 60 giorni, dando quindi al ricorrente la possibilità di un tempestivo ricorso, per vedere se le sue ragioni cautelari siano o meno degne di accoglimento, e così ripristinando una concreta garanzia per il contribuente, pur in rapporto alla necessità di una riscossione più celere e più efficace. È stata anche eliminata una controversa questione riguardante l'efficacia l'efficacia temporale del provvedimento cautelare del giudice, che non è parso alla Commissione potesse sussistere, e anche qui, compatibilmente con le esigenze di bilancio, è stato effettuato un ottimo lavoro, eliminando quel termine. In materia di riscossione dei tributi e dei contributi INPS sono stati poi riallungati una serie di termini. In tema fiscale, naturalmente, una pagina importante è stata quella relativa alla questione dell'Abruzzo: è stata prorogata la sospensione degli adempimenti tributari di imprenditori e lavoratori autonomi nelle zone colpite dal terremoto. La sospensione, finanziata con un aumento delle accise sui tabacchi, non vale per le banche e per le assicurazioni. Forse, anche nel corso del prosieguo in Aula, si potrà fare ancora meglio, come si è letto. Noi ce lo auguriamo, ma ovviamente tutto deve essere compatibile con i saldi. Con riferimento all'aggiornamento del catasto, le modifiche apportate sono finalizzate in particolare ad assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e a disciplinare l'attività dei Comuni e dell'Agenzia del territorio. A lungo si è discusso di questo: vi è stato anche un provvedimento in materia di federalismo fiscale, riguardante, appunto, gli immobili. Riteniamo che questa norma, se ben applicata, potrà dare un significativo apporto alla riduzione dell'evasione fiscale in questo comparto e, quindi, ad una migliore perequazione per tutti i cittadini e ad un aumento del gettito per lo Stato e per gli enti destinatari delle risorse.

Importanti sono stati i provvedimenti di semplificazione a carico della pubblica amministrazione per la cosiddetta impresa veloce, affinché con semplici segnalazioni dell'interessato, nell'ambito degli adempimenti connessi all'inizio dell'esercizio di attività imprenditoriali, sia consentita un'immediata possibilità di iniziare tali attività. Infatti, Infatti, è a carico dell'amministrazione competente, entro un breve lasso di tempo, accertare i requisiti e i presupposti per l'inizio dell'attività; dopo tale periodo l'amministrazione potrà intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile. fraintendimenti sulla salvaguardia di alcune questioni ambientali o dei beni culturali, speriamo di scrivere un testo più netto

alle relative amministrazioni di essere molto più rapide ed efficaci. Infatti, non sempre parlare di ambiente o di beni culturali significa che ci si comporti nel migliore dei modi. Riteniamo che la salvaguardia debba essere assoluta, ma proprio per questo facciamo appello anche a quelle amministrazioni affinché vengano incontro alle esigenze delle imprese mai il proprio potere come ostacolo o impedimento al libero esercizio delle attività. In ultimo, segnalo le disposizioni volte a tutelare la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo questo intervento con alcune considerazioni in ordine ai problemi di più ampia portata che abbiamo di fronte a noi. La Commissione consegna all'Assemblea e al Paese una manovra di dimensioni rilevanti: circa 25 miliardi di Nonostante ciò, ci riteniamo soddisfatti, ma crediamo che si debba fare ancora di più e meglio. meglio. La soluzione dei problemi dell'Italia richiede soluzioni strutturali e capacità di visione strategica. Abbiamo già detto all'inizio che si impone il tema della costruzione di una autentica *governance* economica europea. Sul piano interno, occorre affrontare il tema, mai sufficientemente qui discusso rispetto alla sua urgenza, delle riforme strutturali. Qualcosa è stato già fatto in questa manovra; ho già detto in materia di pensioni; altro dobbiamo continuare a fare. È evidente infatti come, in assenza di un incremento della produttività e di un aumento della partecipazione al lavoro, la nostra economia non possa progredire a ritmi soddisfacenti:

Non vi è dubbio - è più che decennale la serie storica che lo evidenzia - che la diminuzione della crescita è associata all'aumento del debito pubblico. La priorità è quindi una sola: aumentare il tasso di sviluppo del Paese, puntando su tutte le risorse che possono essere mobilizzate. Messi i conti pubblici in ordine, cosa che stiamo facendo, la sfida poi sta nell'impostare nel più breve tempo possibile la manovra di politica economico-finanziaria che verifichi come la finanza pubblica possa aiutare la politica industriale. E non posso non citare in questa sede un problema del quale forse poco si è discusso: si sta giocando a Pomigliano una partita fondamentale per la ripresa industriale dell'Italia. Lì, il 66 per cento dei lavoratori ha ritenuto che quell'accordo dovesse essere approvato, e noi riteniamo che, a partire da quell'accordo, possa riaprirsi una strada per lo sviluppo industriale dell'Italia. Non posso non ricordare come, dopo la Germania, il nostro è il Paese manifatturiero più importante in Europa e che la crescita degli ultimi mesi è stata trainata anche per l'Italia dalle esportazioni; restituire all'Italia questa sua grande vocazione di Paese manifatturiero è sfida importante, che a Pomigliano si sta giocando. Il nostro compito, mantenendo il rigore nei conti pubblici, è contribuire soffermarmi su un'ultima questione. Noi sappiamo come in Italia abbiamo una grandissima forza, che è quella del grande risparmio privato e del piccolo debito privato. Sapete che il Governo ha fatto una giusta battaglia, che ha avuto riscontro positivo in Europa, perché questi parametri siano riconosciuti: non certamente per ridurre il rigore sui parametri pubblici, cioè l'indebitamento ed il debito, ma per far leva su quelle due grandi potenzialità, direi su quei due grandi *asset* dell'Italia, il grande risparmio privato e il ridotto debito privato, per poter associare quelle risorse allo sviluppo della nostra Italia. Questo è il punto sul quale merita svolgere una riflessione,

il debito pubblico vada contenuto e, nello stesso tempo, le risorse private vadano fatte confluire per lo sviluppo industriale.

c'è una forte preoccupazione da parte nostra nel constatare che questa manovra finanziaria, con la blindatura annunciata tramite fiducia, non fa che riproporre in modo acritico e per niente convincente quanto il Governo sta cercando di sostenere davanti al Paese in modo disordinato, confuso e contraddittorio, necessaria coniuga rigore e crescita, è in linea con le richieste dell'Europa e serve al Paese per riportare i conti in ordine e rendere la ripresa duratura. Con le nostre argomentazioni e con le nostre proposte, presentate in Commissione e ripresentate in Aula, dimostreremo invece che questa manovra, già nata male perché iniqua nella distribuzione dei tagli di spesa ed errata nella quantificazione delle voci di entrata, è sprofondata in una confusione non solo tecnica, al punto da superare, con l'emendamento sull'invalidità, i limiti della decenza, non solo economica, perché la tesi secondo cui le politiche di bilancio restrittive bloccano la speculazione è priva di qualsiasi fondamento, ma soprattutto di tenuta sociale, nel trasmettere coscientemente al Paese il pericoloso messaggio che i conti pubblici vengono risanati colpendo gli spreconi e i fannulloni, ossia le autonomie locali ed il pubblico impiego. Contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, la necessità di adottare questa manovra economica non nasce dalla grave crisi finanziaria che ha colpito l'area euro con il drammatico *default* della Grecia ma, in buona sostanza, dall'esigenza di mettere finalmente ordine nei conti pubblici, esigenza sostenuta già dal novembre 2009, quando l'Ecofin, con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, aveva sollecitato l'Italia a mettere in atto, entro il 2 giugno 2010, provvedimenti utili a correggere i saldi di finanza pubblica e porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo. Il Governo quindi, pur negandolo, era ben consapevole già da tempo di questa necessità, a tal punto che nella sua Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica dell'aprile 2010 afferma che, stando fermi gli obiettivi programmatici di indebitamento netto al 2,7 per cento per il 2011, il mantenimento di tali obiettivi richiede una manovra correttiva sul saldo primario pari, in termini cumulati, a circa 1,6 punti percentuali di PIL nel biennio 2011-2012. La realtà dei fatti recenti è nota a tutti: il Governo ha continuato a dirci per mesi che la crisi era superata, che siamo uno dei Paesi che sta meglio, che in fondo sarebbe potuto andare anche peggio. Al riguardo, sono molto significative le considerazioni della Banca d'Italia: "La politica economica ha limitato il danno in una misura stimabile in due punti di PIL, attribuibili per circa un punto alla politica monetaria, per mezzo punto agli stabilizzatori automatici inclusi nel bilancio pubblico e per il resto alle semplici misure di ricomposizione di entrate e spese decise dal Governo". Cerchiamo di capirci ancora meglio: nel 2009 e nel 2010, complessivamente, il Governo italiano ha speso come stimoli alla ripresa, senza dover destinare, come hanno fatto altri Paesi europei, risorse al salvataggio di istituti di credito e senza riforme strutturali,

Noi e non solo noi, visto l'esito dell'incontro con le Regioni, comprese anche quelle virtuose del Nord, riteniamo che la grandissima crisi economica globale e la connessa crisi della zona euro non si risolveranno attraverso tagli ai salari, alle pensioni, allo stato sociale, all'istruzione, alla ricerca, alla cultura e ai servizi pubblici essenziali né attraverso un aumento diretto o indiretto dei carichi fiscali sul lavoro e sulle fasce sociali più deboli. Se per un Governo non c'è atto politico più costitutivo di una finanziaria, se questa finanziaria viene presentata da Tremonti come l'ultima linea da apporre agli attacchi speculativi e alla credibilità internazionale e se su oltre 2.500 emendamenti la metà è stata un'espressione della stessa maggioranza di centrodestra (dai condoni edilizia a quelli delle quote latte), allora vi è il segno tangibile di una conduzione della manovra che ha rivelato insipienze, errori e incapacità. Prima ancora di questioni sul tempo e sul quanto, sarebbero state prioritarie due scelte di fondo, del tutto assenti anche solo a livello di intenzioni nelle proposte del Governo. La ricerca della stabilità dei mercati non può che passare attraverso la ripresa della crescita; il che significa affrontare i motivi del *deficit* di competitività di cui il nostro Paese, più ancora del resto dell'Europa, soffriva già prima della grande crisi e che però ora è diventato evidente ed esplosivo. A livello europeo - su questo sono d'accordo con il presidente Azzollini - il passaggio ineludibile è quello delle priorità in tema di nuove regole e nuovi sistemi di vigilanza e controllo in materia di mercati finanziari che riguardano le banche, gli intermediari sistemici, i sistemi di *rating* e le contrattazioni finanziarie. Mettiamola così, anche perché l'Europa giudica il *quantum* e non il *modus*: questa è una manovra che vuole far cassa nel più breve tempo possibile, non preoccupandosi di ottenere risparmi duraturi e di pensare alla crescita; vorrebbe rassicurare i mercati, ma rischia di dare un'immagine di un Paese alla canna del gas. Qual è il punto di partenza del nostro Paese? I dati di Banca d'Italia, ISTAT ed EUROSTAT consentono di tracciare un primo, ma significativo bilancio dell'attività dei Governi Berlusconi. I principali risultati di queste tre inchieste sono: 430 miliardi di debito pubblico in più, pari a 1.000 euro per ogni cittadino italiano per ciascun anno in cui Berlusconi ha governato (quindi, 7.500 euro per ciascuno di noi); una minore crescita del PIL rispetto ai principali Paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Germania), pari quasi a un punto per ogni anno sotto la piena responsabilità dei suoi Esecutivi, equivalenti a una perdita di circa 60 miliardi di euro in cinque anni; un tasso di crescita della spesa pubblica negli anni di Governo berlusconiano pari al 3,7 per cento l'anno, quasi il doppio della crescita dei prezzi, che è del 2 per cento in media l'anno. In tutte e tre gli aspetti considerati, i Governi italiani di centrodestra si sono dimostrati i peggiori d'Europa. Il provvedimento al nostro esame, signor Presidente, dichiara di basarsi principalmente su riduzioni e razionalizzazioni di spesa, ma ha in termini di stabilizzazione dei conti pubblici il difetto di avere un carattere essenzialmente emergenziale. La gran parte dei tagli proviene da misure di congelamento della spesa (il blocco dei salari pubblici), di riduzione al margine, come i molti tagli orizzontali, o di semplice dilazione di pagamento, come nel caso delle liquidazioni dei dipendenti statali. Sono, invece, sostanzialmente assenti gli interventi strutturali sulle dinamiche della spesa. Negli ultimi dieci anni la spesa pubblica è crescita in media del 4,6 per cento l'anno e la parte più consistente è rappresentata dai consumi intermedi della pubblica amministrazione, cresciuti anche in assenza di scelte esplicite in tal senso dei Governi, al punto da assorbire tutti i risparmi di spesa per interessi prodotti dall'adesione all'euro. La manovra non dà alcuna risposta convincente al problema e senza interventi strutturali, capaci di correggere i meccanismi di produzione della spesa e di mettere in discussione abusi consolidati e pratiche clientelari diffuse lungo tutta la Penisola con varia intensità, i proclami dell'attuale manovra rischiano di essere ancora una volta smentiti. La correzione imposta dalla manovra non serve, dunque, come si fa credere, a migliorare gli obiettivi, ma a raggiungerli. La finanza pubblica, nonostante quanto ripetutamente affermato dal Governo, non è affatto sotto controllo. L'avanzo primario, pari al 3,5 per cento del PIL nel 2007, è precipitato a -0,6 per cento in due anni è stato peggiorato di oltre quattro punti (oltre 62 miliardi di euro). Ed ancora, la manovra avrà effetti depressivi sull'economia e l'occupazione. Non può fare a meno di ammetterlo lo stesso Governo con la Nota di aggiornamento alla relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, presentata in Commissione bilancio al Senato. Il decreto-legge targato Tremonti avrà un impatto negativo sulla crescita economica pari allo 0,5 per cento del PIL nel triennio 2010-2012. Se il cuore della manovra, dunque, è tutto nel blocco delle retribuzioni del pubblico impiego, nel taglio dei fondi ai Comuni e alle Regioni (complessivamente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pensionamento, per la chiusura delle finestre, che frutterà altri 6,5 miliardi, allora è evidente, signor Presidente, che pagano il conto i ceti popolari e brindano gli speculatori e gli evasori. Mettiamola così: la speculazione finanziaria che ha provocato la crisi attuale si è fatta, per così dire, rifinanziare e garantire dagli Stati sovrani che a loro volta recuperano con dure manovre antisociali che rendono ancora più gravi e insostenibili le disuguaglianze del nostro Paese. contesta la necessità di intervenire per correggere i conti pubblici, anche se lo si fa per colpa di una politica economica del Governo che ha sbagliato le previsioni, sottovalutato la crisi, rinviato le soluzioni per mancanza di una strategia, ricercato una fiducia nascondendo le verità e non proponendo politiche di bilancio che fossero equilibrate e sostenibili agli occhi di tutti: delle famiglie, la cui fiducia è fondamentale per la crescita, e delle imprese, che devono essere sempre pronte per preparare l'avvenire. Senza se e senza ma non è accettabile una manovra di tagli pesanti fatti senza equità, senza pensare allo sviluppo, all'innovazione, all'occupazione. Pagano i lavoratori pubblici e della scuola e anche del settore privato; pagano i lavoratori in mobilità che solo in parte potranno andare in pensione senza incappare nella finestra mobile; pagano i cittadini, perché 10 miliardi tolti a Regioni e Comuni avranno come conseguenza un taglio ai servizi e alle persone. Già con il taglio lineare del 10 per cento delle missioni di spesa di ciascun Ministero nell'ambito delle spese rimodulabili, se si considera quanto avvenuto nel passato, ossia il fatto che il decremento della spesa ha riguardato in larga parte le spese in conto capitale, inevitabilmente verrà ridotta la parte più importante per lo sviluppo poiché i Ministeri non avranno risorse necessarie per finanziare gli investimenti e anche molte risorse destinate alle politiche sociali. Ma non basta. Il Governo di fatto, con i tagli imposti, preclude l'esercizio di molte delle funzioni di competenza regionale, di assoluta sensibilità sociale ed economica, oltre a qualsiasi azione anticiclica e di sviluppo del territorio. ciò avviene in una fase di preoccupante deterioramento dei rapporti tra il Governo e le Regioni che non ricorda precedenti nel passato. Non è solo una guerra di numeri: il contributo cumulato regionale, secondo gli stessi governatori, sarebbe di 8,6 miliardi su 36, pari al 23,8 rispetto al combinato disposto dei tagli dello Stato quantificati in 12,7 miliardi su 84 miliardi di spesa discrezionale, ossia soltanto il 15,1 Ma restano irrisolti due grandi problemi. Il primo è una possibile ulteriore aggressione all'ammontare dei fondi FAS destinati alle Regioni, compromettendo pesantemente l'intero impianto programmatorio previsto dal quadro strategico nazionale 2007‑2013, approvato con decisione dalla Commissione europea. Il secondo è che solo dieci piani attuativi regionali hanno avuto la presa d'atto del CIPE, mentre gli ulteriori dieci attendono da quasi un anno di essere iscritti all'ordine del giorno. Va poi detto che alla delibera CIPE non è seguito alcun trasferimento di risorse per le Regioni che ne avevano comunque maturato il diritto. Il fondo per il Servizio sanitario nazionale contribuisce alla manovra per 1,2 miliardi di euro, di cui circa la metà rappresenta tagli al personale. Tra contratti e convenzioni saranno bloccati per tre anni aumenti per 1,7 miliardi. Effetti devastanti si prospettano dal blocco del *turnover*. Un taglio micidiale, che comporterà la perdita di 78.000 unità da qui al 2014. Un esercito. Meno personale, meno servizi. Per i lavoratori del settore pubblico, dopo la sottostima delle risorse previste dalla finanziaria 2010 per il rinnovo dei contratti, ora si prevede che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non possa superare quello del 2010. Per il lavoro privato i sacrifici si sostanziano nel rinvio dell'accesso al pensionamento, attraverso l'introduzione della cosiddetta finestra a scorrimento. Sulla questione del Mezzogiorno dobbiamo riconoscere che c'è almeno un po' di pudore nel parlare di fiscalità di vantaggio, mentre nella delega sul federalismo si parlava di fiscalità di sviluppo. È difficile, infatti, pensare che le Regioni del Mezzogiorno, tanto più dopo i tagli previsti dalla manovra in discussione e, per alcune di esse, l'obbligo di far ricorso alla leva fiscale per coprire i disavanzi sanitari, abbiano risorse per avviare una concorrenza fiscale nei confronti delle altre aree per attirare nuove iniziative. E anche quando si ritenesse che una concorrenza fiscale tra Regioni è possibile, è tutto da vedere se, data la situazione di arretratezza, la carenza di infrastrutture, il degrado istituzionale e l'esposizione alla malavita organizzata, in cui molte zone delle Regioni interessate dalla fiscalità di vantaggio si trovano, sia sufficiente far credere che la riduzione virtuale, soltanto virtuale, dell'IRAP possa compensare la forbice del divario tra Nord e Sud. Per non parlare poi della norma fantascientifica finalizzata ad attirare in Italia imprese di altri Paesi europei. A queste imprese verrebbe, infatti, riconosciuta la possibilità di scegliere la normativa fiscale più favorevole fra le 27 esistenti all'interno dell'Unione. Non solo non si capisce come possa essere concretamente applicabile, ma appare in palese contrasto con le regole comunitarie e con la Costituzione italiana. italiana. Signor Presidente, piuttosto che assegnare patenti di cialtroneria, il Governo dovrebbe, una volta per tutte, assumersi la responsabilità di intervenire con la definizione di un progetto Mezzogiorno, che miri a migliorare la quantità e la qualità della spesa dei fondi straordinari, individuando con chiarezza poche priorità condivise e concentrando risorse vere. È uno sforzo necessario, una prova di maturità della classe dirigente del Mezzogiorno e dell'intero Paese. La manovra governativa realizzata con questo decreto-legge è stata presentata dal Governo come una pietra miliare nella lotta all'evasione fiscale. Va detto che è positivo che il Governo su molti aspetti abbia deciso, almeno a parole, di fare un passo indietro, abbandonando le guerre ideologiche e le ricette a base di slogan che lo avevano portato ad abrogare molte delle disposizioni introdotte dal Governo Prodi. In numerosi ambiti il passo indietro è clamoroso: dopo aver abrogato il registro clienti e fornitori, viene introdotto un seppur parziale obbligo di comunicazione elettronica delle fatture; viene reintrodotto, dopo averlo cancellato con squilli di fanfare, un limite massimo ai pagamenti in contanti; vengono inserite norme su specifiche questioni come le imprese apri e chiudi e quelle in perdita sistemica, su cui si era già concentrata l'attenzione negli anni passati, quando l'attuale maggioranza, allora opposizione, gridava alla vessazione dei contribuenti. Tirando le somme, però, su 7 principali provvedimenti antievasivi che dovrebbero portare 4,4 miliardi nel 2011, per almeno 5 sussistono dei forti dubbi. Si salvavano la preclusione alla compensazione da parte dei contribuenti in presenza di ruoli definitivi non pagati, che vale secondo la relazione tecnica 700 milioni di euro, e il potenziamento dei processi di riscossione, del valore stimato di 400 milioni di euro. E diciamo "si salvavano" prima che avvenisse l'intervento della Confindustria. Questo significa che circa i tre quarti della portata effettiva della manovra antievasione, appaiono, se non proprio scritti sulla carta, di certo in un forte dubbio di evanescenza. La prima cosa da fare, signor Presidente, è sbarazzare il campo dall'equivoco che le cose, dopo tutto, non vanno poi così male. Nella fase di crisi, il nostro reddito è calato più della media Unione europea (il Le previsioni per il 2010-2011 non indicano che la ripresa italiana sarà più rapida degli altri Paesi dell'area euro. quasi un giovane su tre è disoccupato ed è importante acquisire piena consapevolezza di questo fatto, di un'intera generazione vittima di questa crisi, per uscire dal mondo di favola in cui si è cercato di far vivere negli ultimi due anni il nostro Paese. Certo, si dirà che i dati OCSE pongono la disoccupazione, a maggio in Italia, attestata all'8,7 per cento, vale a dire un incremento di 2 punti percentuali dall'inizio della crisi, inferiore alla crescita media degli altri Paesi nello stesso periodo. Peccato che si ometta di riferire la seconda parte del rapporto OCSE in cui si rileva che la ripresa dell'attività economica non porterà a una creazione significativa di occupazione nel breve periodo e che i salari italiani sono agli ultimi posti tra i Paesi avanzati; dietro di noi ci sono solo la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Corea, la Grecia e la Spagna. In secondo luogo, bisogna evitare di illudersi: vi sono almeno tre ragioni per cui la questione della crescita non può più essere rimandata. C'è, prima di tutto, un rallentamento ormai ventennale del tasso di crescita della produttività. La seconda ragione è che la scarsa crescita della produttività si traduce in bassi salari e mortifica il potere d'acquisto delle famiglie. Il terzo motivo è che soltanto attraverso una crescita sostenuta del reddito è possibile ridurre il peso del nostro debito pubblico senza compromettere eccessivamente la capacità di spesa dello Stato. L'Italia dei Valori, con gli emendamenti presentati alla manovra, ha voluto proporre una vera e propria contromanovra rispetto a quella predisposta dal Governo. Le nostre proposte intendono non solo contribuire alla riduzione del debito ma soprattutto promuovere lo sviluppo e sostenere le fasce più deboli. Abbiamo predisposto un pacchetto di emendamenti che costituiscono una manovra biennale di 65 miliardi di euro di cui 33 miliardi dedicati alla riduzione del *deficit* e 32 miliardi allo sviluppo, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale a lavoratori e piccole e medie imprese. Le nostre proposte emendative si sono sviluppate soprattutto su tre direttrici: risanamento, con particolare riferimento al contrasto all'evasione fiscale e contributiva e all'adozione di alcune misure a carattere fiscale; equità; crescita. Ogni intervento di riduzione ragionieristica dei *deficit* dei bilanci pubblici nazionali, signor Presidente, noi riteniamo sarebbe inutile se non fosse accompagnato da riforme strutturali per rilanciare la crescita, sostenere la domanda interna, la nostra capacità di competere sui mercati internazionali dei Paesi emergenti con la qualità dei nostri prodotti, che accompagnino il nostro sistema produttivo verso una riconversione ecologica del nostro modello di sviluppo e della nostra società. Nulla di tutto ciò è avvenuto in questa manovra finanziaria. Basta vedere l'ultimo ritocco subito da questa manovra, che con l'articolo 49 fa saltare tutta la normativa di tutela ambientale e il regime delle autorizzazioni in vigore da sempre in Italia, cancellando con un colpo di spugna l'articolo 9 della Costituzione e il codice dei beni culturali, varato proprio dal Governo Berlusconi. Noi proponiamo una manovra anticiclica, pari a quasi 4 punti di PIL per il biennio 2011-2012, che riduca la pressione fiscale, trasferendola almeno in parte dal lavoro, dalle famiglie, dalle imprese alla rendita speculativa. Riteniamo urgente che le azioni dei mercati vengano regolamentate e che la speculazione finanziaria sia fortemente ridimensionata. Elenco le misure nel dettaglio. Proponiamo l'addizionale del 7,5 per cento sui capitali regolarizzati tramite lo scudo fiscale; il ripristino delle norme di contrasto all'evasione fiscale introdotte dal Governo Prodi; il recupero immediato delle somme dovute dai contribuenti che hanno aderito al condono fiscale 2003-2004 e che non hanno pagato buona parte delle rate, secondo quanto già da tempo denunciato dalla Corte dei conti; la tassazione con l'aliquota del 20 per cento delle plusvalenze finanziarie speculative, con l'esclusione dei rendimenti dei titoli di Stato; il ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale e la reintroduzione dell'ICI su determinate categorie catastali, quali le case di lusso; la messa all'asta delle frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre, come hanno fatto altri Paesi (gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia). Per le banche, chiediamo la riduzione della quota di deducibilità per le sofferenze creditizie dallo 0,30 allo 0,20 per cento. Per i veri tagli ai costi della politica, proponiamo: la soppressione parziale delle Province, in attesa della eliminazione nella nostra Costituzione dell'istituzione Provincia; l'eliminazione del vitalizio per i parlamentari nazionali e per i consiglieri regionali, includendo in tale misura anche gli ex parlamentari e gli ex consiglieri regionali; nuove regole per gli appalti e per l'intervento della Protezione civile, nonché per combattere la corruzione. Per operare veri tagli alla spesa pubblica, proponiamo: una riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni, attraverso un taglio modulabile, soprattutto a carico delle amministrazioni centrali, e il rafforzamento del ruolo della CONSIP; la riduzione delle spese militari; la soppressione dei finanziamenti previsti per il ponte sullo Stretto di Messina; la soppressione di tutti gli enti inutili (secondo la lista di Padoa-Schioppa ce ne sono 119). A favore dei cittadini, dei lavoratori, delle famiglie, anche al fine di sostenere la domanda interna, abbiamo proposto: gli aumenti delle detrazioni per carichi familiari; l'alleggerimento del carico IRPEF sui redditi bassi e medi da lavoro e da pensione, diminuendo l'imposta sulle tredicesime e attraverso il meccanismo delle detrazioni; la garanzia degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici. Per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese, abbiamo previsto la riduzione del costo del lavoro nell'imponibile IRAP per le piccole e medie imprese e il pagamento dell'IVA al momento in cui si incassa e non in anticipo.

ma è una necessità, soprattutto nel momento in cui il tema centrale diventa quello di estirpare la piaga dell'evasione fiscale. nella sostanziale equità dell'intervento pubblico, è improbabile che si attivi un'opinione pubblica decisa a mettere all'angolo gli evasori fiscali e a fare sacrifici comuni. La seconda questione riguarda il pesante indebolimento che ha subito il concetto di solidarietà all'interno del sistema italiano, in questi ultimi anni. Se passa il concetto del ciascuno per sé e Dio per tutti, si fa fatica a mantenere la coesione e senza coesione non c'è la possibilità di vincere la sfida dello sviluppo a livello di Nazione. Il Paese, oggi più che mai, ha bisogno di uno scatto di responsabilità solidale, a fronte di una crisi che non è più di tanto congiunturale, perché rimette in discussione il modello di sviluppo per il futuro. abbiamo tutti onestà intellettuale nel valutare, sapere e riconoscere che se questo è il *quantum* e il *modus* di tale manovra, da qui a otto mesi saremo di nuovo a ragionare di manovre correttive dei conti pubblici. Se infatti il problema è - com'è anche - quello di riassorbire il disavanzo pubblico, gli strumenti che si intendono attivare non potranno raggiungere lo scopo e, nel migliore dei casi, sposteranno soltanto nel tempo la soluzione del già grave problema del debito pubblico. Se inoltre il problema è - com'è anche - quello del debito pubblico, esso non può essere affrontato indirettamente con le manovre di riduzione dei *deficit* annuali, nella speranza - perché in fondo tale resta - che il reddito cresca, che cresca il settore manifatturiero e con esso il gettito tributario. Signor Presidente, concludo richiamando una riflessione. C'è qualcuno che dice che l'esperienza è la capacità di fare errori nuovi non potendo più ripetere quelli vecchi. Noi dell'Italia dei Valori, con le nostre proposte, faremo di tutto, in Aula e fuori, per convincere gli italiani che questa esperienza del Governo non può più esercitarsi sulla vita e sul futuro del nostro Paese. *(Applausi

minoranza*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la debolezza più grave della manovra è la sua mancanza di ambizione e di coraggio. La crisi può sempre costituire un'occasione per migliorare i fondamentali del Paese, per affrontare quelle riforme strutturali che in condizioni normali sono più difficili da realizzare; un'occasione che non doveva essere sprecata.

di fronte ad un'urgenza ostinatamente negata per un lungo periodo. Vi sarebbe stato lo spazio per un discorso franco al Paese. Certamente sarebbe stato possibile fare appello alle migliori energie della Nazione costruire un consenso reale attorno alle cose che servono. Ce lo saremmo aspettato, l'opinione pubblica avrebbe capito il senso di sacrifici necessari per il bene comune, purché equamente ripartiti e finalizzati a lasciare un Paese migliore, più giusto e più competitivo. Il Presidente del Consiglio ha scelto un'altra strada, prima negando l'emergenza, poi mettendosi sulla strada di chi vuol dividere più che unire: sembra che non sappia governare se non lavorando per dividere l'opinione pubblica e sconquassare ogni rapporto istituzionale e politico, per dividere la sua stessa maggioranza, che ormai occupa gli spazi della comunicazione per i litigi permanenti, le minacce, e non per le decisioni. La scelta dello scontro permanente, dunque, a cominciare da quel perentorio «se fosse al Governo la sinistra saremmo come la Grecia» pronunciato dal Presidente del Consiglio. Vedete, colleghi, anche nella più aspra delle contese politiche c'è un debito con la verità. Presidente del Consiglio che fa questa affermazione è un signore che ha governato l'Italia per 10 degli ultimi 16 anni. Egli ha ricevuto in eredità un Paese il cui debito era al 103,5 per cento del PIL e lo ha portato quest'anno al 118 per cento, appunto il livello della Grecia. Eletto sulla promessa "meno tasse per tutti", ha portato la pressione fiscale alrecord storico del 43,2 per cento, coltivando in ogni occasione l'invito alla slealtà fiscale; quest'anno, per la prima volta dopo 19 anni, viene azzerato l'avanzo primario, che è il risparmio necessario per poter abbattere il debito. Egli ha soprattutto indebolito la competitività del Paese. L'annuale classifica del *World Economic Forum* ha registrato negli anni di governo dell'Ulivo un avanzamento da parte dell'Italia di 13 posti nella classifica mondiale per la competitività, frutto di politiche concrete di liberalizzazioni, di aperture di mercati, di riforme portate a compimento. Negli anni in cui ha governato Berlusconi,

Questi sono i dati. Questi sono i fatti. Gli insulti non li possono nascondere. Noi però preferiamo parlare d'altro. Vogliamo guardare al futuro; vogliamo pensare ai problemi reali del Paese. Siamo un Paese che da troppo tempo cresce troppo poco: nei dieci anni antecedenti la crisi, il PIL italiano è cresciuto di 15 punti, rispetto ai 25 punti della media euro. Siamo un Paese che perde produttività: la produttività del lavoro negli ultimi 10 anni è cresciuta del 3 per cento rispetto ad una media dell'area euro di 14 punti. Bassa crescita affidata a scarsi investimenti e a bassi salari: ed infatti siamo agli ultimi posti in Europa per il livello dei salari, e nell'ultimo biennio si è registrato un calo di quasi il 20 per cento per gli investimenti fissi nell'industria. La produttività totale dei fattori per il settore manifatturiero arretra di 5 punti rispetto al 1995, mentre la Germania ne guadagna 30 e la Francia 26. Una parte della popolazione rischia di restare esclusa dal circuito della produzione; la partecipazione delle donne al lavoro è tra le più basse in Europa; drammatica è la condizione giovanile: il 79 per cento dei posti di lavoro persi nell'ultimo periodo riguardano giovani tra i 18 e i 29 anni. La disoccupazione giovanile è al 29,5 per cento. Ci sono in Italia 2 milioni di giovani che non studiano, non lavorano, non cercano neppure lavoro. L'Italia è un Paese in cui aumentano le diseguaglianze. Nella classifica OCSE l'Italia è il secondo Paese europeo come ampiezza nella distribuzione della diseguaglianza della ricchezza e il primo Paese per immobilismo sociale: non c'è quasi più ascensore sociale; chi nasce nella parte bassa della scala sociale ha una elevata probabilità di restarvi. Nel 2000, secondo il test OCSE-PISA i nostri studenti dimostravano una capacità superiore alla media comunitaria: vi era solo un 19 per cento di studenti con scarsa capacità di lettura. Dopo meno di dieci anni la percentuale è andata ben al di sopra della media europea, raggiungendo il 27 per cento quasi un terzo dei giovani italiani non sa procurarsi informazioni da un testo scritto, capirne la logica interna e metterlo in relazione con le nozioni che già possiede. La demografia continua a restare fuori da un discorso politico pubblico. Eppure abbiamo dei problemi particolari: siamo il Paese più vecchio d'Europa; l'indice sintetico che misura il rapporto tra popolazione anziana e popolazione giovane supera il 30 (sei punti sopra la media europea); in cinque anni è più che raddoppiata la presenza di cittadini stranieri, e sono stati anni di bassa crescita economica. Si preferisce parlare di sicurezza invece che di politiche rigorose, di una necessaria integrazione. È questa un'analisi troppo pessimistica? No, è un'analisi realistica. Non siamo pessimisti. Anzi, pensiamo che l'Italia abbia le risorse anche per vincere questa sfida. danno il meglio di sé di fronte alle difficoltà, con la ricchezza di uno spirito imprenditoriale diffuso, un capitale sociale ancora molto forte, punti di eccellenza che restano competitivi. Non abbiamo avuto le bolle speculative che hanno caratterizzato altre economie; il sistema bancario si è dimostrato solido; vi è un risparmio privato che compensa abbondantemente lo stato del debito pubblico; abbiamo una base manifatturiera che pochi Paesi occidentali hanno. Solo che gli italiani, le nostre imprese non possono più farcela da soli. Hanno bisogno che la politica faccia la propria parte, decidendo con lungimiranza, promuovendo le riforme necessarie ad abbattere barriere e rendite inattaccabili, per recuperare e organizzare la forza strutturale del Paese, quella che si trova nell'economia reale. Così com'è questa manovra non corrisponde a queste esigenze. Abbiamo cercato di dimostrare che è possibile cambiarla, mantenendo un quadro di rigore finanziario in direzione di una maggiore equità e di una maggiore attenzione alla crescita. I nostri emendamenti sono in campo. Ancora una volta il Presidente del Consiglio ha dichiarato che l'opposizione «produce una raffica di no su tutto senza che ci venga fatta una proposta alternativa». Veramente in queste settimane i no senza motivazione, senza controproposte, sono stati quelli del Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi. L'opposizione ha messo in campo invece una propria proposta alternativa basata su tre pilastri. Intanto il fisco. La crisi è l'occasione per reimpostare la struttura fiscale italiana verso una maggiore equità. Ricordo che negli ultimi 30 anni i redditi da lavoro dipendente sul valore aggiunto sono scesi dal 66 al 53 per cento, ma il peso dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sul lavoro dipendente è balzato dal 52 al 70 troppo pochi pagano troppe tasse. Finalmente vi siete convinti che la lotta all'evasione fiscale è un elemento indispensabile. Avete detto: dalle persone e dalle imprese alle cose. Bene, noi proponiamo di incominciare a farlo. Almeno un euro su due di quelli provenienti dalla lotta all'evasione fiscale secondo la nostra proposta deve andare ad alleggerire la posizione dei contribuenti onesti. Un fisco amico della famiglia, avete detto molte volte. Si può incominciare a farlo. Abbiamo proposto dì raddoppiare le detrazioni per figli aumentando la soglia di detraibilità, ferma da molti anni. Oppure, di rendere deducibili le spese per *baby-sitter*, asili nido, badanti, che condizionano pesantemente i bilanci delle famiglie. Oppure, iniziare ad agire con uno strumento universale, la dote fiscale per i figli, prevedendo un assegno di 3.000 euro annui fino al diciottesimo anno di età. Aiuti concreti, dunque. Scegliamo, scegliete, ma qualcosa va fatto. Per le imprese, proponiamo di togliere il costo del lavoro dall'imponibile IRAP delle piccole imprese e dei professionisti. Avete detto che avreste cancellato l'IRAP. Incominciamo a fare qualcosa. Con l'operazione cuneo fiscale fu tagliato da noi circa un quarto dell'IRAP; oggi si può fare un altro passo in avanti in un momento di grande *stress* per il sistema delle piccole imprese. Diciamo che il finanziamento di queste misure di alleggerimento fiscale può trovare copertura attraverso due misure. Una sovrattassa di 3 punti sui capitali regolarizzati attraverso lo scudo fiscale, ricordando che nessun Paese europeo che abbia fatto operazioni analoghe ha usato un'aliquota così bassa per la regolarizzazione e che, al contrario di quanto affermato dal Governo e come era ovvio, solo una minima parte dei capitali scudati si sono tradotti in investimenti sul sistema Italia. Una seconda azione riguarda l'avvio di una tassazione più equa delle rendite finanziarie. L'aliquota attuale al 12,5 per cento non ha riscontro tra i maggiori Paesi europei ed è particolarmente iniqua rispetto alla tassazione dei redditi di lavoro e di impresa. ne propone perciò l'innalzamento al 20 per cento, escludendo da questo aumento i titoli di Stato. Infine, appare urgente un intervento sulla fiscalità della casa, con una tassazione secca al 20 per cento dei redditi da affitto, accompagnata da una detrazione del 20 per cento delle spese di affitto per gli inquilini, un provvedimento all'inizio costoso, ma che rapidamente si farà pagare da solo, con una forte emersione del nero, realizzando un vantaggio sia per i piccoli proprietari, con una maggiore convenienza per l'investimento immobiliare, sia sotto il profilo di un sostegno del reddito per le famiglie di inquilini. Il secondo pilastro è la spesa pubblica. Va ridotta la spesa corrente improduttiva, ma non è pensabile agire senza strumenti razionali e con un così forte squilibrio tra centro e periferia: il sistema delle autonomie locali dovrebbe contribuire con 14,8 miliardi di euro, i Ministeri solo con 3,4 miliardi Negli ultimi cinque anni, in verità, la spesa della pubblica amministrazione centrale è aumentata di 1,2 punti rispetto al PIL, mentre per Comuni e Regioni al netto della spesa sanitaria il peso è diminuito di due decimi di punto. Lo Stato che non sa controllare la propria spesa scarica sulla periferia le proprie inadempienze. Il Governo non ha saputo costruire un patto concordato con il sistema delle autonomie, come lo richiederebbero la Costituzione e la nuova legge di contabilità. Così si sta profilando un federalismo di cartapesta in cui i costi *standard* saranno solo una esercitazione statistica; i Comuni dovranno far fronte ai tagli dello Stato centrale incapace di controllare la propria spesa con un aumento della pressione fiscale; le Regioni, secondo le uniche promesse fatte dal Governo, potranno continuare a sfondare la spesa sanitaria per sprechi e non per migliori servizi senza alcuna reale sanzione. Non è possibile intervenire così. Noi proponiamo un'altra strada: un contributo più rigoroso di razionalizzazione della spesa corrente, con l'introduzione di una norma programmatica generale che agisca sull'intero bilancio dello Stato e non solo sulle quote cosiddette rimodulabili. quello di tagliare la spesa di due punti percentuali per il primo biennio e poi di contenerla entro il 50 per cento della crescita del PIL nominale. Questo è l'obiettivo per una maggiore disciplina di bilancio. Lo strumento è completare per tutti i Ministeri l'analisi della spesa compiuta dalla Commissione per la finanza pubblica, purtroppo destituita dal vostro Governo, che per i 4 Ministeri che aveva esaminato aveva dimostrato la possibilità di introdurre azioni amministrative innovative con il risparmio di qualche miliardo di euro. Proponiamo poi una serie di azioni che darebbero risultati rilevanti: l'unificazione dei due grandi enti previdenziali INPS e INPDAP; la razionalizzazione e la riduzione della struttura periferica dei Ministeri; l'introduzione della ricetta e del fascicolo elettronico per contrastare gli abusi della spesa farmaceutica; una drastica riduzione dell'uso delle auto blu e dei voli di Stato; un prosciugamento delle ipertrofiche strutture della Presidenza del Consiglio; l'attuazione concreta della valutazione dell'efficienza della pubblica amministrazione e il premio del merito, che avete promesso, tradotto in una norma di legge ed ora colpevolmente abbandonato. Tutte cose concrete che si possono fare, riequilibrando la manovra a favore di Regioni e Comuni, secondo principi di merito e di efficienza, costruendo insieme obiettivi rigorosi di rientro dall'eccesso di spesa. Infine, vi è il terzo pilastro: misure per lo sviluppo. I fondi mobilitabili sono certo ridotti e occorre concentrarsi in alcuni settori strategici. Abbiamo proposto che il credito d'imposta per la ricerca e per il Mezzogiorno vada liberato dalla famigerata esperienza del *click day*. Non si può affidare ad una lotteria il sostegno ad investimenti strategici per lo sviluppo. si sostiene la *green economy*; in Italia si fa l'esatto contrario eliminando i benefici per l'efficientamento energetico degli edifici e alterando il regime delle incentivazioni per le fonti rinnovabili, compromettendo investimenti già programmati. Sul piano delle infrastrutturazioni abbiamo sottolineato in particolare la necessità di procedere con la realizzazione della banda larga, che può trovare sostegno dai fondi che possono derivare da una rapida vendita delle frequenze rese libere dal digitale terrestre, e la necessità di un intervento urgente sulla portualità. È indispensabile agire sul Patto di stabilità interno almeno per le politiche di investimento, liberando energie finanziarie disponibili che rapidamente si trasferirebbero sulla domanda di opere pubbliche. Sempre per lo sviluppo proponiamo un piano straordinario di interventi a sostegno dell'autonomia finanziaria per le giovani generazioni e misure fiscali per incentivare il lavoro femminile. Se non si mobilitano le tre grandi risorse inespresse, Mezzogiorno, giovani e donne, è improbabile riacquistare un sufficiente ritmo di crescita. Tra le proposte per lo sviluppo avanziamo alternative ai tagli indifferenziati per la cultura, la scuola, la ricerca. Fattori strategici per la crescita, investimenti in capitale umano, che è l'unica materia prima che possiede il Paese: non capire questo significa avere gli occhi chiusi sul futuro. Proponete ai giovani una mini naja di tre settimane. Una perdita di tempo che costa allo Stato 20 milioni di euro. Non sapete trovare questa somma per i giovani ricercatori che costruiscono il futuro della competitività italiana. Mini naja, non ricerca, non università. *(Applausi dai abbiamo proposto liberalizzazioni e semplificazioni, che significano risparmi ingenti per le imprese ed innalzamento della produttività del sistema Paese, in particolare per i mercati dell'energia, le banche, le assicurazioni, i farmaci. L'efficacia di questi interventi è dimostrata dai dati: il mercato dell'elettricità, più liberalizzato di quello del gas, ha avuto *performance* di prezzo molto migliori per i consumatori. Una parzialissima liberalizzazione nel settore dei farmaci, con le lenzuolate Bersani, ha comportato per il consumatore un ribasso dei prezzi del 5 Siamo convinti che si debba semplificare il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione. Vi abbiamo fatto proposte più incisive di quelle da voi approvate. Con paletti essenziali, però: le imprese devono avere un quadro dì certezza del diritto, troppe norme si sovrappongono in modo confuso. Quando sono in gioco beni pubblici indisponibili come quelli ambientali, paesaggistici e monumentali occorre impedire manomissioni irreversibili. Occorre che i controlli *ex post* siano rigorosi, continui, efficaci e le sanzioni pesanti, altrimenti ancora una volta sarebbero i disonesti a fare la concorrenza sleale agli onesti. Parlate di modificare l'articolo 41 della Costituzione, che invece giustamente afferma la natura sociale dell'impresa, ma intanto andate in direzione opposta. Se ci sono parole estranee allo spirito della manovra queste sono concorrenza e mercato. Infatti agite ancora una volta intervenendo in modo casuale sulla filiera del farmaco, senza riguardo per le imprese che investono, senza rompere le situazioni di monopolio e di profitto ingiustificato, senza agire sui macroscopici conflitti di interesse. Intervenite sul mercato dell'energia appropriandovi di una parte di potenziali risparmi che spetterebbero ai consumatori: una vera nuova tassa sull'energia. Tassate le riserve delle assicurazioni, che sono sostanzialmente dei debiti e, in un mercato chiuso, sono costi che si trasferiranno sul consumatore. Vi ostinate a premiare 67 imprese agricole che non vogliono pagare le multe per le quote latte sforate, in un settore in cui sono in corso processi per truffa, penalizzando tutto il resto del mondo agricolo ed esponendo l'Italia a sanzioni comunitarie che saranno pagate da tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo dimostrato che se si volesse si potrebbe fare una manovra con ben altro respiro. Per questo insistiamo: la parte sbagliata della manovra non è il presunto rigore. Presunto, perché una parte delle entrate sono sovrastimate e una parte dei tagli di spesa non si realizzeranno. Presunto, perché in Commissione avete peggiorato la manovra, con relazioni tecniche sui costi degli emendamenti spesso del tutto inattendibili. La parte sbagliata non è il rigore, è la sua mancanza di ambizione, la rinuncia a combattere per rendere più competitivo il sistema Italia. Italia. Signor Presidente, quando nel 1932 Franklin Delano Roosevelt lanciò la prospettiva politica del *New Deal* seppe prendere in mano una nazione prostrata dal fallimento di una economia avida e speculativa ed avviarla ad un nuovo slancio. Ricordava Roosevelt in quel famoso discorso: «I leader repubblicani non solo hanno fallito nel concreto, ma hanno dato la prova di non possedere una prospettiva nazionale, poiché nel momento del disastro essi non hanno avanzato nessuna speranza, non hanno indicato alcuna strada alla gente per tornare ai luoghi della sicurezza e della salvezza del nostro modo Concludeva Roosevelt: «Io impegno voi tutti, impegno me stesso a un *New Deal* con il popolo americano. Proclamiamoci tutti profeti di un nuovo ordine di competenza e coraggio». le elezioni su queste parole di speranza. La storia si ripete. Anche oggi ci vorrebbero, appunto, competenza e coraggio. Queste doti sono richieste alla politica particolarmente nei momenti di crisi. E' ciò che manca alla manovra che avete proposto. La mancanza di coraggio è dimostrata anche dall'intenzione, già annunciata informalmente, di porre l'ennesima questione di fiducia. Mancanza di coraggio nell'affrontare nel merito le contraddizioni della maggioranza e con argomenti di merito le proposte dell'opposizione. Vogliamo togliere ogni alibi a questa scelta. Il gruppo del Partito Democratico è disponibile a ridurre a 25 il numero degli emendamenti da discutere in Aula. Sono quelli che configurano la manovra che ho illustrato; 25 emendamenti, signor Presidente. Abbia il coraggio la maggioranza di giudicarli di fronte all'opinione pubblica e di spiegare i motivi dell'eventuale diniego. Direte di no? È l'ennesima prova della stanchezza di un Governo che non corrisponde più agli interessi generali e che ha perso l'autorevolezza necessaria a guidare il Paese.

Nel corso di una maxioperazione mista, tra Carabinieri e Polizia, che ha coinvolto ben tre procure, Reggio Calabria, Milano e Monza, sono stati effettuati 300 arresti e, nell'ambito di essi, sarebbe sarebbe stato arrestato il numero uno della 'ndrangheta calabrese, Domenico Oppedisano. Ritengo di interpretare questo applauso, da me pienamente condiviso, come il senso di compiacimento e ringraziamento per le attività svolte dalle forze dell'ordine, dalla magistratura e anche dal Ministero degli interni per questa importantissima operazione, che dà il segnale che lo Stato c'è,

che attiene forse ad una questione settoriale, ormai divenuta di scarsa rilevanza - sia per quanto riguarda l'attenzione del Governo sia per quanto riguarda tutti gli organi di cosiddetta informazione

ma anche una misura che, pur nella sua settorialità, è altamente significativa, discriminatoria e particolarmente odiosa. Questo comma

6 aprile 2009 vedono prorogate al 15 dicembre le disposizioni in tema di sospensione del pagamento delle tasse,

perché questa differenziazione della disciplina di proroga, per esempio, per tipologia di reddito, non si giustifica da alcun punto di vista. Questa norma dice che i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore ai 200.000 euro vedono prorogato al 15 dicembre il pagamento delle tasse; gli altri pagano dal 1° luglio.

posto un po' d'ordine per quanto riguarda il recupero del gettito fiscale del 2009, che invece di essere recuperato in cinque anni sarà spalmato sui prossimi dieci. colleghi, che nel maxiemendamento è prevista, su sollecitazione di tutti, un'altra proposta, quella della zona franca. Molto bene. Ma, detto tutto questo, in in un Paese dove l'evasione fiscale forse è la vera piaga, e giustamente gli organi di informazione in questi giorni ci hanno raccontato che ville e *yacht* appartengono a nullatenenti,

sarà poco - che sia un buon messaggio quello di dire ai terremotati dell'Aquila che dal 1° luglio alcuni di loro ricominceranno a pagare le tasse? Con questa modalità e con questa forma?

tralascio le procedure, su cui tornerò dopo - con il famoso «progetto case»; gli altri stanno ancora tutti negli alberghi o sfollati presso parenti. Ma di quale attività produttiva stiamo parlando?

su cosa è successo nella cosiddetta e tanto sbandierata ricostruzione dell'Aquila, ma chiunque abbia messo piede in quella città sa perfettamente che di progetti seri di ricostruzione non si vede l'ombra, che quella è e continua ad essere una città fantasma, che la gestione emergenziale della Protezione civile ha forse avuto più di una lacuna,

la gestione emergenziale affidata alla Protezione civile e di restituire agli enti preposti la pienezza delle competenze, individuando fonti certe di copertura finanziaria e assicurando forme di coinvolgimento decisionale della popolazione locale. Tutto questo abbiamo voluto dire anche presentando un ordine del giorno che, grazie alla fiducia così come annunciata dagli organi di stampa, evidentemente decadrà e non sarà discusso. Rimane quindi, di tutto quello di cui si dovrebbe discutere nella manovra, questa parte, che è di per sé, ripeto, non solo settoriale, ma significativa per tutto quel che indica e perché implica una disparità di trattamento rispetto ad articoli della Costituzione e, alla luce della non ricostruzione, è particolarmente odiosa oltreché discriminatoria tra i cittadini dell'Aquila. Non la farò lunga, però credo che le manifestazioni di questi giorni dicano molto della delusione seguita a promesse mirabolanti di ricostruzioni in tempo record,

né la *governance*: non si vede alcunché. Per tutti questi motivi, per violazione di articoli della Costituzione, ed in particolare degli

le proposte accettate dal Governo che ho citato poc'anzi non risolvano, non sanino, non aiutino, non adeguino all'entità e alle

non certo per distrazione ma per una precisa scelta politica, perché è noto a tutti che abbiamo sin dall'inizio affermato che questa manovra era necessaria al Paese per mantenere gli impegni nei confronti dell'Europa e dei mercati, pur avendo, sempre dall'inizio e poi via via accentuando ancor di più il nostro giudizio, contestato nel merito il il contenuto della manovra stessa. Lo abbiamo fatto in Commissione per più di un mese, presentando proposte precise di miglioramento e proposte alternative

Pur tuttavia, il tema posto dalla senatrice Bonino è molto rilevante. È stato, peraltro, uno degli argomenti principali che hanno occupato la discussione in Commissione. Nel merito giuridico, costituzionale e fattuale, la questione posta dalla presidente Bonino è fondata, perché, contrariamente a ciò che si dice sulla stampa e a ciò che ha detto il presidente relatore Azzollini, pur con la sua completa, ampia e, come come sempre, puntuale relazione, non c'è stata e non c'è la sospensione di tasse, imposte e contributi per i cittadini dell'Aquila e del cratere dal 1° luglio fino a dicembre. C'è una parzialissima sospensione,

fino a 200.000 euro. Quindi per i rilievi costituzionali relativi alla disparità di trattamento tra i contribuenti, alla violazione del principio della capacità contributiva (anche tenendo conto del fatto che con 200.000 euro di volume di affari si può avere un percettore di reddito alto o un percettore di reddito zero,

Più in generale, il tema della fiscalità - signor Presidente, lei lo sa bene, avendo con molta cortesia accolto e ascoltato una delegazione capeggiata dal sindaco dell'Aquila e composta rappresentanti istituzionali, della società civile e delle organizzazioni economiche e sindacali del cratere del sisma abruzzese ‑ è stato gravemente sottovalutato dal Governo. Lo è stato nel passato e lo è tutt'oggi. Con ogni probabilità su di esso bisognerà tornare. La sospensione, che in altri eventi sismici era stata disposta per un periodo oscillante all'incirca tra i 20 e i questo caso è stata di fatto quasi integralmente bloccata a 15 mesi, pur in presenza di un terremoto molto più grave degli altri.

la rateizzazione è partita molti anni dopo: addirittura 10 o 12 anni dopo), per 10 anni ulteriori al 40, al 20 o al 10 C'è questo annuncio positivo del Governo di accrescere le rate da 5 a 10 anni, ma non è sufficiente. Da gennaio, signor Presidente, tutti i cittadini e tutti i contribuenti pagheranno -

Non sarebbe giusto, purtuttavia, tacere - e in tal senso procederemo nel corso della discussione con gli interventi degli altri colleghi - alcuni risultati positivi che noi abbiamo ottenuto Mi riferisco al fatto che la zona franca urbana, già prevista nel decreto terremoto, che era stata degradata a zona a burocrazia zero nel testo originario del decreto, è stata ripristinata in virtù di un emendamento a prima firma del presidente Marini, ma con il sostegno attivo di tutti i colleghi abruzzesi, di maggioranza e di opposizione.

Ecco perché, signor Presidente, la fondatezza e la rilevanza della questione posta dalla collega Bonino. Il rischio che le popolazioni interessate - che sono esasperate, e lo sono giustamente - non comprendano la posizione di contrarietà a tale questione induce molti di noi a votare a favore, pur lasciando il nostro Gruppo piena libertà di voto, per le ragioni di carattere generale cui mi sono riferito all'inizio del

presentata obiettivamente debole e del tutto infondata. Gli interventi, poi, sono andati nel merito della questione abruzzese, ma qui siamo in una sede in cui bisogna parlare soltanto dell'aspetto costituzionale. le posizioni dei cittadini si differenziano fra quelle di coloro che godono di un reddito autonomo, professionale o di impresa, e quelle di coloro che sono impiegati o lavoratori comunque subordinati, differenziando il trattamento si viola l'articolo 3 Noi sappiamo che tale articolo si riferisce a situazioni eguali o omogenee e quando si va a violare una di queste situazioni, omogenee, si mette in essere o un trattamento non costituzionalmente conforme o un trattamento irrazionale e, come tale, anch'esso non costituzionalmente conforme. Qui però è evidente che il diverso trattamento dei lavoratori in proprio, autonomi e imprenditori, si basa sul concetto di aleatorietà dei proventi. Mentre i lavoratori subordinati continuano ad avere il loro compenso, i lavoratori non subordinati rischiano quotidianamente in proprio e, in una situazione come quella dell'Aquila, in cui non si è ancora ripresa la vita normale, il loro rischio è tangibile. Di qui la conclusione che questa diversificazione non sia lesiva dell'articolo 3 della Costituzione e che la scrittura da parte del Governo Mi pare poi che richiamare, su queste basi, l'articolo 53 non abbia alcun significato: non siamo in una logica di capacità contributiva e di progressività. D'altro canto, se proprio volessimo, anche per completezza, guardare all'articolo 53, leggeremmo che: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Ma in questo caso non ci troviamo in una situazione normale, per cui le capacità contributive devono essere stimate e messe in un'ottica di progressione. La situazione di fatto a mio avviso prescinde dall'articolo 53, per cui, a fronte di redditi diversi, alcuni dei quali fortemente aleatori, il legislatore ha messo in essere correttamente questa normativa.

di compatibilità costituzionale, ma con una serie di appunti sulle norme che presentavano aspetti problematici.

con la previsione di più controlli, che sono certamente utili e giustificati. Lamentavamo che il nuovo regime degli avvisi di accertamento dell'impugnazione per sospensiva davanti alle commissioni tributarie ripristinasse addirittura il principio negativo del *solve et repete* e prefigurasse la violazione dell'articolo 24, cioè della difesa del cittadino, perché concedendo solo 150 giorni

porta a zone a burocrazia zero e a destinare le risorse per le ex zone franche ai

Il fatto che all'Aquila sia stata ricostituita la zona franca urbana ci fa sperare anche per le zone franche urbane del del Centro e del Nord, che non sono state considerate alla stregua di quelle del Sud. Qual è il problema oggi? non c'è ancora un decreto attuativo che porti le zone franche urbane residue ad ottenere i finanziamenti già stabiliti

che opera in Italia, ma soltanto quando sia la prima volta che questo intervento si realizza. Anche questo era uno dei punti che avevamo evidenziato. Non posso soffermarmi a lungo su altri aspetti. Vorrei solo dire che l'esame della 1a Commissione è stato estremamente attento, che la Commissione bilancio - che ringrazio, nel suo presidente, senatore Azzollini, ed in tutti i suoi membri - ha fatto tesoro anche delle nostre osservazioni, e che quindi credo che questa manovra, così necessaria, come ha spiegato il senatore Legnini, e risolta da noi in questo modo

2 verserebbe in stato di evidente incostituzionalità). Mi pare che il gioco non valga la candela; quindi, non solo sul piano giuridico ma anche sul piano sostanziale, chiedo che la richiesta della senatrice Bonino venga respinta.

il Paese sta attraversando un momento particolarmente difficile per l'economia, l'occupazione, le condizioni di vita e di lavoro di molte famiglie, la competitività del sistema Paese, lo stato dell'etica pubblica, le prospettive della crescita. Ne è una riprova anche questa manovra, a cui siamo chiamati certo per il rispetto di impegni sollecitati a scala europea, per fronteggiare meglio le tensioni dei mercati, il rischio di aggressione alle economie dei Paesi più vulnerabili dell'eurozona, così da tutelare la stabilità dell'euro e l'equilibrio sistemico. Ma in questa manovra c'è una zavorra che non si può imputare al contesto internazionale; le sue ragioni sono tutte interne e discendono dagli errori della politica economica attuata dal Governo in questi due anni. Conosciamo bene la narrazione che avete pervicacemente accreditato, prima negando l'esistenza della crisi, poi minimizzandola, per lasciare successivamente intendere che già ne stavamo uscendo prima e meglio degli altri. Lo avete detto anche a ridosso dell'adozione della manovra, presentata come stato di necessità per non fare come la Grecia e poi, dopo un po' di pudore e di silenzio nel corso di queste settimane, di fronte ai tanti focolai di critica e di protesta, da alcuni giorni il presidente Berlusconi ha ripreso a propinarci la trita novella che le cose stanno andando bene e non c'è ragione di preoccuparsi: si tratta della solita propaganda distruttiva dei comunisti e della stampa di sinistra, Sono balle spaziali, queste! Lo dicono gli stessi documenti governativi. Dalla Relazione sull'economia e la finanza pubblica del maggio 2010, si ricava che la correzione non servirà comunque a migliorare gli obiettivi dei conti pubblici, magari in funzione di sostenere la crescita come sta avvenendo per altri Paesi europei, ma soltanto, e faticosamente (ce lo auguriamo) a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei conti pubblici, perché la nostra finanza pubblica, nonostante quanto ripetutamente affermato dal Governo, è tutt'altro che sotto controllo. In particolare, per quanto riguarda le spese, si segnala che le uscite finali al netto degli interessi sono aumentate di 57 miliardi di euro, di cui 3 miliardi per spese in conto capitale e ben 54 miliardi di spese correnti al netto degli interessi. E anche per il 2010 c'è una crescita che è il risultato del saldo di un incremento grande delle spese correnti e di una riduzione, ancora una volta, degli investimenti. Non ci sono ragioni per ricondurre alla crisi l'impennata della spesa corrente, il conseguente crollo del saldo primario e l'esplosione del *deficit* di bilancio. Anzi, in proposito, sarebbe necessaria una risposta non filosofica, ma documentata responsabilmente, da parte del Ministro dell'economia sull'andamento delle entrate e delle spese, che le entrate sono significativamente inferiori a quanto programmato in precedenti documenti e invece le spese sono assai superiori. Del resto, non possiamo non ricordare che, all'inizio del 2008, quando è terminata l'esperienza del Governo Prodi, i conti pubblici erano sotto controllo e il *deficit* era abbondantemente dentro i parametri comunitari. Sono state le scelte successive, dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa anche per i redditi medio-alti alla vicenda Alitalia e alla cancellazione delle norme antievasione, che hanno pesato sui conti pubblici per diversi miliardi di euro, proprio nel momento in cui si evidenziavano i primi segnali di instabilità economica e finanziaria dei mercati internazionali. La dissipazione di quelle risorse ha spiazzato il Governo proprio nel momento in cui servivano interventi di spesa per affrontare in funzione anticiclica la crisi economica. Così, non avendo a disposizione spazi di manovra per gli interventi veramente necessari, il Governo ha tenuto un atteggiamento di inerzia, difforme dalle scelte adottate dai Governi di altri Paesi che, al contrario, proprio per reagire alla sfida del periodo di crisi economica e dei mercati finanziari, hanno deciso di attuare non solo misure di indirizzo e di sostegno alla loro economia, ma soprattutto di affrontare il nodo di rilevanti riforme strutturali. Per discutere utilmente di quali linee dovessero caratterizzare la manovra di cui ci occupiamo si sarebbe dovuto partire da qui. Questo ragionamento vale a maggior ragione considerando la scelta, che non possiamo non apprezzare, di introdurre nella manovra molte misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Si riconosce, finalmente, l'esistenza di un problema enorme, che è non solo un tema di sostanza morale, ma anche una questione strutturale che indebolisce la competitività e fiacca le energie del Paese. L'evasione fiscale, nel suo complesso, sottrae all'erario più di 100 miliardi di gettito all'anno. Ne vengono, come conseguenza, una alterazione nella parità di concorrenza tra le imprese, con indebiti vantaggi per quelle che evadono rispetto a quelle leali con il fisco, ed effetti distorsivi sulla struttura dei costi. E con la conseguenza di determinare un peso fiscale eccessivo sulla parte dei contribuenti che adempiono il loro dovere fiscale, oltre a minare lo spirito civico del Paese per una neanche troppo nascosta tolleranza che si è tenuta verso i comportamenti illegali. Anche qui una domanda sarebbe più che legittima: quanto ci è costato, in questi due anni, l'azzeramento di quell'insieme di strumenti introdotti nel biennio di Governo 2006-2007 proprio per il contrasto all'evasione? L'effetto sul gettito del complesso di queste azioni fu quantificato dal Governo di allora in circa 23 miliardi di euro (è l'importo di questa manovra), certo anche come riflesso di una significativa inversione, allora, di *compliance* da parte dei contribuenti. Indubbiamente oggi invertire la tendenza sarà difficile, dopo anni di predicazione a favore della banalizzazione e giustificazione dell'evasione fiscale, segnali legislativi che sono stati dati di tolleranza verso l'evasione e l'elusione, di condoni plurimi fino all'ultimo scudo che ha generosamente beneficiato gli evasori che avevano trafugato illegalmente fondi all'estero. Tuttavia, ben vengano

Come le disposizioni sull'obbligo delle fatture telematiche per importi superiori a 3.000 euro, che pure rappresentano un passo avanti nella lotta all'evasione, anche se la soglia resta ancora troppo elevata per costituire un filtro davvero efficace. E così pure vanno bene quelle misure mirate al contrasto dei fenomeni delle imprese "apri e chiudi" e di quelle in perdita "sistemica" e all'incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa. In materia di microevasione si sarebbe forse potuto avere più coraggio anche recuperando il divieto per i professionisti di percepire compensi in contanti entro determinate soglie. Aspettiamo una prossima conversione anche su questo terreno. Resta tuttavia l'incertezza sulle stime circa l'entità del recupero di gettito dalla lotta all'evasione: si tratta di entrate molto incerte nel *quantum* (quale sarà il gettito recuperato dai maggiori controlli? Quanto i maggiori controlli porteranno ad un incremento dell'adesione spontanea? Quanto l'adesione spontanea diminuirà per effetto dei passati e, forse, futuri condoni?), e pertanto sarebbe stato più prudente contabilizzare tali possibili, auspicabili, entrate solo a posteriori, come aveva fatto più correttamente lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze nella scorsa legislatura. L'aspetto da incentivare nella lotta all'evasione è quello non dell'estemporaneità, ma della fedeltà fiscale, che passa necessariamente attraverso la certezza della fine dei condoni. In questo quadro, sarebbe risultato un segno davvero di forte discontinuità - e avrebbe dato credibilità a tutto l'impianto - se la maggioranza avesse accolto tra i nostri emendamenti quelli in cui si proponeva un prelievo aggiuntivo sui fondi rimpatriati da chi ha beneficiato dello scudo fiscale a un costo di regolarizzazione che è un decimo di quanto è stato previsto negli altri Paesi. Oltretutto, più del 50 per cento di costoro ha mantenuto quei fondi all'estero, evitando di farli rientrare nel circuito a sostegno dell'economia nazionale, come si voleva far credere da parte del ministro Tremonti. Insieme a quella misura avevamo proposto l'inasprimento dei prelievi nei confronti di coloro che, ad oggi, dopo sette anni, non hanno finora ottemperato ai versamenti dovuti per il condono del 2003, e poi l'adozione di più incisive disposizioni per il contrasto all'elusione fiscale. Da ultimo, una sottolineatura, che riprendeva già il collega Giaretta nel suo intervento per illustrare la relazione di minoranza, su un aspetto che è clamorosamente omesso e che accresce i profili di iniquità di questa manovra. Se si ipotizza che possano essere recuperati quasi 8 miliardi di euro dal contrasto all'evasione e all'elusione, non è accettabile che una quota significativa degli stessi, almeno la metà, non sia destinata alla riduzione della pressione fiscale a favore delle categorie che rispettano gli obblighi contributivi e impositivi. Altrimenti, il risultato sarà, come è, quello di un ulteriore aumento della pressione fiscale. Bisogna iniziare a spostare il peso fiscale da imprese e famiglie alle rendite, e contribuire per questa via a ridurre l'eccesso di disparità nella distribuzione del reddito e del carico fiscale. Per questo abbiamo proposto alcune misure, che venivano già richiamate e che cito solo per titoli: un'azione di riduzione della pressione fiscale su tutte le donne lavoratrici (sarebbe un elemento dinamico di sviluppo per l'occupazione e la crescita della ricchezza del Paese); una serie una serie di interventi a favore delle famiglie, con un sistema di sostegno mediante gli assegni per i figli (un *bonus* di 3.000 euro che cresca gradualmente con l'estendersi della possibilità di disporre di maggiori risorse), un sistema di detrazioni per le spese di educazione, di assistenza, ivi incluse le spese per le cosiddette badanti, un sistema di interventi che aumenti le detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che è fermo da ormai quindici anni. Interventi concreti che insieme con quelli verso le imprese - di esenzione dall'IRAP per la parte del lavoro e di tassazione forfettaria, per dare un sollievo alle microimprese che più stanno risentendo delle conseguenze della crisi - possano in qualche modo aiutare a reggere questo passaggio difficile. un intervento di fiscalità sulla casa, con la cedolare secca e l'aiuto agli inquilini, una misura che ha il valore virtuoso di far emergere il sommerso e di creare le condizioni di incentivazione di un mercato altrimenti stagnante. Risulta necessario inoltre affrontare - e mi avvio a concludere, Presidente - la questione indifferibile della tassazione delle rendite finanziarie, che registra tuttora in Italia una percentuale non in linea con gli altri Paesi europei, determinando in questo modo un elemento di freno che costituisce (poiché in qualche modo è distorsivo nell'allocazione del risparmio) un elemento che accentua le ragioni della bassa competitività del sistema economico italiano. infine sottolineare che è indispensabile (ormai non vorremmo più sentire solo parole ed evocazioni mediatiche) affrontare il tema di una riforma organica della materia fiscale. C'è l'esigenza di intervenire con misure correttive volte a riequilibrare il sistema di imposizione con l'obiettivo di correggere, in un'ottica di maggiore equità, la distribuzione della ricchezza nel Paese, che è fortemente diseguale. Bisogna che su questo tema si ragioni seriamente smettendola di usare il mantra del federalismo fiscale come la panacea di tutti i mali, grazie a cui ci sono risorse per tutti e si possono ottenere rilevanti risparmi, anche nuove tasse che, accorpando quelle esistenti, moltiplicherebbero le risorse da introitare. Prima o poi questo gioco delle tre carte dovrebbe veramente finire e dovremmo cominciare a diventare un Paese che discute seriamente di tali temi. Anche perché - e concludo - voi nelle more dell'IMU, l'imposta municipale unica, e dei decreti che verranno il federalismo lo avete azzoppato sul nascere con i tagli che proponete con questa manovra. Soprattutto, così facendo, avete mortificato le aspettative di molti cittadini di cui continuate a carpire la fiducia e che però molto presto vi cominceranno a presentare il conto. Signor Presidente, onorevole Giorgetti, presidente Azzollini, colleghi, ogni sostantivo ha necessità di avere degli aggettivi per essere meglio esplicitato, e allora questa manovra che noi ci accingiamo a votare ha necessità di essere ulteriormente spiegata. Immaginando di dover utilizzare degli aggettivi, mi sono interrogato rispetto all'effettivo dolore che provoca

come obiettivo il conseguimento della ripresa del nostro Paese. La riduzione lineare della spesa applicata ai vari Ministeri, ai trasferimenti alle Regioni, ai Comuni, alle Province e agli enti locali avvia per davvero, anche con la riduzione e la razionalizzazione degli enti pubblici, la riduzione dei costi della politica. Un esempio valga per tutti: l'ipotesi di sradicare dal Ministero dello sviluppo economico le stazioni sperimentali per affidarle alle camere di commercio. Questo è un esempio emblematico che offre la mia Regione, la Campania,

periodo l'amministrazione potrà solo intervenire in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile. Inoltre, abbiamo autorizzato il Governo a regolamentare la materia al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese.

l'aumento salariale alla produttività e all'efficienza delle imprese. Un altro tema centrale è quello del Mezzogiorno, l'area del Paese che presenta la maggiore potenzialità di crescita rispetto alla produttività. Al riguardo va ricordato

possa per davvero avviare una rivoluzione in questa direzione e creare le condizioni affinché questo Mezzogiorno possa effettivamente decollare. Ecco perché altrettanto positiva è la previsione della fiscalità di vantaggio

la norma che consente alle imprese europee di operare in Italia scegliendo di mantenere, in alternativa a quello vigente nel nostro Paese, il regime fiscale del Paese

vi sono ampi margini per incrementare la garanzia di spazi minimi di concorrenza, anche grazie allo strumento della legge annuale a ciò deputata. Vi sono spazi per una maggiore semplificazione burocratica a favore delle imprese.

la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi. In particolare, si stabilisce che nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio,

A proposito del Mezzogiorno ho idee molto precise. Nel Mezzogiorno d'Italia bisogna smetterla con la sindrome del risarcimento, immaginando di avere un credito. Certo, abbiamo un credito;

Gran parte di essi sono volti ad accertare quali benefici di natura economica e fiscale, a quale titolo e di quale entità vengono erogati (fondi, contributi ed elargizioni di vario genere) alle associazioni animaliste e ambientaliste, che nel nostro Paese sono più di 45: un numero sproporzionato rispetto al resto dell'Europa. Alcune di esse hanno bilanci da capogiro e conti economici più simili a società per azioni che ad ONLUS e *non profit*. Esprimo il mio profondo rammarico come parlamentare e come esponente della maggioranza nel vedere mortificato il mio impegno e annuncio fin da ora che eserciterò tutte le mie prerogative istituzionali per vedere pienamente rispettate le mie aspirazioni.

ai quali sono stati promessi mari e monti, ma che invece versano in gravi difficoltà economiche e psicologiche. Mi scrive Adelisa Pitti: «Ieri mi ha telefonato l'impiegata di una società di recupero crediti, per conto di Sky. Mi dice che risulto morosa dal mese di settembre del 2009. Mi chiede come mai. Le dico che dal 4 aprile dello scorso anno ho lasciato la mia casa e non vi ho più fatto ritorno. Causa terremoto. Il *decoder* Sky giace schiacciato sotto il peso di una parete crollata. Ammutolisce. Quindi si scusa (...). Poi, premurosa, mi chiede se ora, dopo un anno, è tutto a posto.

Poi mi invita a raccontarle cosa è la mia città oggi. Ed io lo faccio». Le chiedo scusa, signor Presidente, se utilizzerò ancora 30 secondi per concludere il mio intervento. «Le racconto del centro militarizzato. Le racconto che non posso andare a casa mia quando voglio. Le racconto che, però, i ladri ci vanno indisturbati. Le racconto dei palazzi lasciati lì a morire. Le racconto dei soldi che non ci sono, per ricostruire. E che non ci sono neanche per aiutare Le racconto che torneremo a pagare le tasse ed i contributi, anche se non lavoriamo. Le racconto che pagheremo l'ICI ed i mutui sulle case distrutte. E ripartiranno regolarmente i pagamenti dei prestiti. Anche per chi non ha più nulla.

Che lo Stato non versa ai cittadini senza casa, che si gestiscono da soli (ben 27.000), neanche quel piccolo contributo di 200 euro mensili che dovrebbe aiutarli a pagare un affitto.

I giornali, però, i giornalisti, la televisione, la stampa di regime questi fatti non li raccontano. Per questo, signor Presidente, le chiedo di sollecitare il Governo a venire a rispondere in quest'Aula.